Capigruppo del 2 ottobre e comunicati ai Gruppi. Le risoluzioni sulla Nota di aggiornamento dovranno essere presentate entro le ore 10. Eventuali emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro 30 minuti dal momento dell'espressione del parere del Governo.

che ha colpito i mercati internazionali; in secondo luogo, risulta decisivo il rafforzamento molto rilevante dell'euro in rapporto al dollaro. Ritengo che queste cause dovrebbero essere indagate a fondo; tuttavia gli obiettivi di finanza pubblica per il nostro Paese rimangono invariati. *(Brusìo)*.

svolge egregiamente il suo dovere. L'indebitamento netto che nel 2006, con la relazione previsionale e programmatica, era stato cifrato

il decreto approvato a giugno che, come noto, utilizzando una quota dell'extragettito, ha prodotto un'iniziativa di redistribuzione sociale e di sostegno ai finanziamenti (in particolare, alle Ferrovie dello Stato e all'ANAS). In ogni caso, va ricordato che c'è un miglioramento del 2007 sul 2006 di 0,7 punti percentuali: credo si tratti di un dato molto significativo, che va ascritto alle azioni di politica economica del Governo.

Migliorano le previsioni tendenziali del *deficit*: la spiegazione sta nel fatto che il fabbisogno del settore statale, cifrato in 25 miliardi, è inferiore di 11 miliardi rispetto al 2006.

un ragionamento che credo sia necessario ribadire anche in Aula. L'opposizione sostiene che se non ci fosse stato il decreto di giugno e se non ci fosse il decreto di accompagnamento alla finanziaria che esamineremo nei prossimi giorni, il *deficit* sarebbe stato più basso rispetto a quanto certificato dalla Nota di aggiornamento.

la questione della copertura della finanziaria per il 2008, essa non deriva da riduzioni di spese ma dall'utilizzo delle maggiori entrate che, anche nel 2008, dovrebbero riprodursi. Intanto, voglio ricordare che sono previsti, come copertura della finanziaria che esamineremo nei prossimi giorni, 4,6 miliardi

nei prossimi mesi. Voglio ricordare, in particolare all'opposizione, che nei cinque anni di Governo del centro-destra, la spesa è aumentata di 2,5 punti percentuali.

Mi auguro, Presidente, che venga presentata nei prossimi giorni la relazione che certifica quanta parte dell'extragettito derivi

ci può aiutare a comprendere meglio le iniziative che devono essere adottate nel prossimo futuro. Al riguardo insisto e mi auguro che il Governo presenti questa relazione nei prossimi giorni. Infine, Presidente, segnalazioni che ritengo positive. Con questa Nota di aggiornamento viene certificato l'aumento dell'avanzo primario che, nei cinque anni di Governo precedente, era arrivato a zero, adesso siamo sopra il 2 per cento. Quindi, con l'aumento dell'avanzo primario, abbiamo finalmente la ripresa della diminuzione dello *stock* del debito pubblico. l'andamento della pressione fiscale, essa è certamente alta, ma viene stabilizzata e, ovviamente, noi ci auguriamo si adottino tutte le iniziative per ridurla nei prossimi anni. Infine, vi è il rallentamento dell'aumento della spesa in rapporto al PIL che viene anche questa stabilizzata. L'obiettivo, come dicevo, è quello di ridurla, di renderla più efficiente, di spendere meglio. La scommessa del prossimo futuro è aumentare la produttività del settore pubblico,

Grazie, senatore Ripamonti, per questa integrazione utile per la discussione.

palesemente scoperti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Vorrei chiedere se ci sono state indicazioni dal parte della Presidenza della Repubblica. La seconda informazione

che ha formalmente dichiarato nel corso dei mesi e delle settimane scorse un extragettito stimato in 25 miliardi di euro, come mai questi 25 miliardi di extragettito, rispetto al dato tuttora vigente di entrate di 703 miliardi nella Nota di aggiornamento che stiamo discutendo... PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore

avendo lo stesso dichiarato 25 miliardi complessivi di extragettito rispetto al dato di dicembre, perché nella Nota di aggiornamento al DPEF ne mette solo 19 e perché

prego. la Nota di aggiornamento al DPEF, nel precedere la finanziaria, aggiorna il quadro macroeconomico previsto a luglio, quindi qualche mese prima, alla luce dei recenti avvenimenti internazionali e nazionali. Ora, nella relazione che accompagna la Nota si rivedono le stime del DPEF a causa della recente crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti, la la crisi finanziaria che ha fatto parlare tutte le prime pagine dei giornali, riguardante i mutui immobiliari, i cosiddetti mutui facili, che non hanno retto all'incremento dei tassi a migliaia di contraenti che non hanno più potuto restituire i ratei dei mutui. Conseguentemente sono saltate le banche e sono stati polverizzati milioni di risparmiatori che avevano acquistato i titoli obbligazionari di quelle banche. Ebbene, rispetto a questa motivazione non siamo d'accordo. Il ministro Tommaso Padoa-Schioppa ha più volte dichiarato che il nostro sistema bancario è rimasto stabile rispetto al mercato immobiliare. Pertanto, situazioni come quelle registrate negli Stati Uniti hanno avuto una portata molto limitata, tale da non influire sul nostro sistema finanziario. Una domanda è d'obbligo: perché allora rivedere le stime del DPEF di luglio? La lettura che facciamo non è molto più realistica

perché tiene conto da una parte delle stime non veritiere del DPEF e dall'altra di eventi non desiderati, come l' onerosità dell'accordo sul *welfare* che tanto sta facendo discutere all' interno del centro-sinistra. Qualcuno ha provato a giustificare, molto più intelligentemente del ministro Padoa-Schioppa, la ricaduta nazionale della crisi finanziaria statunitense con l'apprezzamento ad 1,42 dell'euro, a seguito del taglio di 50 punti base del tasso di sconto da parte della Federal Reserve, come faceva notare il relatore di maggioranza. Il ragionamento fatto è stato il seguente: la stima della crescita del PIL al 2008 si è basata sugli andamenti tendenziali dei consumi interni e del positivo recupero dell'*export*; la svalutazione del dollaro favorisce una migliore penetrazione commerciale della produzione USA rispetto a quella europea e italiana determinando una crisi recessiva di queste economie. Come giustamente ha fatto notare al sottoscritto il sottosegretario Sartor nel dibattito di ieri in Commissione, l'*export* italiano sta subendo una contrazione di volumi ma non di valore, stante la *performance* del sistema produttivo più esposto all'internazionalizzazione che in questi anni ha saputo ristrutturarsi sul lato dell'innovazione di prodotto, che rappresenta la strada competitiva più idonea per penetrare i mercati esteri. Sicché non si ha una contrazione della bilancia dei pagamenti e non si ha una flessione del PIL nella componente dell'*export*. Se è vera questa analisi rimane la componente macro dei consumi interni che tende a contrarsi, determinando una riparametrazione degli obiettivi di crescita. Questo dato, che la nota in discussione ci offre, conferma la mia tesi e quella dell'opposizione che la politica del Governo Prodi, tesa ad aumentare la pressione fiscale, avrebbe sottratto all'economia italiana quote di reddito significative, determinando una fase recessiva proprio mentre l'economia mondiale ed europea cresceva. Oggi, infatti, gli italiani sono più poveri del 2006, perché se nel 2006 milioni di italiani non arrivavano alla quarta settimana del mese, adesso non arrivano alla terza settimana. I dati dell'Agenzia delle entrate commentati qualche giorno fa dal collega Eufemi nel dibattito sull'assestamento dimostrano che la media dell'aumento delle addizionali comunali, che il centro‑destra aveva congelato, è del 30 e che le addizionali regionali si stabilizzano intorno al 17 per cento di media. Pertanto, se con la finanziaria 2007 avete vantato per i redditi sotto i 40.000 euro lordi un modesto vantaggio fiscale, nel ridisegnare la curva distributiva dell'IRPEF, con i bilanci di Regioni e Comuni, vi siete rimangiati tutto. Anzi, avete morso pure quello che avevano lasciato come disponibilità di reddito, con la riduzione delle aliquote marginali dell'IRPEF, i governanti del centro-destra. Se poi immaginiamo che, accanto alla contrazione dei redditi a causa della pressione fiscale, che nel 2008 toccherà il livello del 1997, quando l'Italia entrò all'euro, cioè il 43 per cento, ben 2 punti in più del 2006; se ci mettiamo anche l'aumento dei prezzi di prodotti di prima necessità, come pasta, pane, latte e trasporto pubblico, ben si comprende la condizione in cui versa il Paese oggi. Nonostante questa evidenza, continuate ancora a ripetere la bugia di Visco e del Governo che le norme tributarie approvate con i due decreti di Visco servono a combattere l'evasione fiscale. Sfugge ai faziosi e a coloro che sono in malafede che l'aumento della pressione fiscale si ha quando aumentano le tasse a coloro che già le pagano. Se fosse vero che i provvedimenti di rigore fiscale adottati da Visco e da questa maggioranza di centro-sinistra avessero avuto una qualche efficacia, oggi registreremo un aumento di gettito delle entrate così rilevante, senza aumento in verticale della pressione fiscale ma, al contrario, una diminuzione della stessa pressione a causa dell'allargamento della platea dei contribuenti, grazie al recupero dell'evasione. Niente di tutto questo è accaduto o sta accadendo. Si ha l'extragettito o "tesoretti", come li chiamate voi, perché è aumentato il carico fiscale di chi già paga le tasse, di chi è già contribuente. Questo è ormai nella coscienza degli italiani - a ragione - il Governo delle tasse. Che sia così è dimostrato da un altro dato fornito dalla Guardia di finanza: nel 2007 sono stati compiuti meno recuperi di evasione del 2006. Sicché anche la lotta all'evasione ed elusione con i gendarmi non sta funzionando. Non solo: anche se funzionasse, tutti sanno che il rapporto tra il pagato e l'accertato è di dieci a cento, in un arco di tempo che va da sette a State quindi sbagliando tutto e gli errori li stanno pagando gli italiani, così come dimostrate anche con questa Nota di aggiornamento. Alcuni dati sono eloquenti. Rispetto alle previsioni del Documento di programmazione cento, scende all' 1,9 e quello previsto per il 2008 all'1,9 scende all'1,5-1,6 per cento. L'indebitamento previsto per il 2008 al meno 2,5 per cento, con l'inglobamento degli effetti incrementali dell'uso del "tesoretto" con il decreto-legge n. passa al 2, 2 per cento. Tale dato è previsto come tendenziale, però a legislazione vigente; non sconta, cioè, gli impegni già sottoscritti, le prassi consolidate ed eventuali nuove iniziative che nella tabella XIII.13 del DPEF erano cifrate in 21 miliardi, perché si diceva in tale sede che gli oneri sarebbero stati pagati attraverso la riduzione di spesa ossia il famoso *spending review*; invece, in questa Nota leggiamo che il saldo netto da finanziare, ossia la differenza tra entrate finali e spese finali dello Stato, sarà incrementato di 10 miliardi, passando dai previsti 24 miliardi a 34. si incrementa a causa dell'incameramento, nel debito dello Stato, del debito delle Regioni nel settore sanitario. Quindi, si diceva: niente manovra. In sostanza, dicevate: lasciateci utilizzare il "tesoretto" perché l'economia tira meglio del previsto; non metteremo più tasse per il futuro. I buoni propositi sono smentiti dalla manovra economica di 10 miliardi e 900 milioni che proponete per la finanziaria. In due mesi vi siete anche qui rimangiato tutto. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, con un'ultima considerazione. Con le parole e Con le parole e i buoni propositi di questa maggioranza non si fa buona politica, così come hanno dimostrato con l'inattuazione del comma 507 della finanziaria 2007 sui tagli di spesa, così come hanno dimostrato di non saper trasformare in norme le pur lodevoli analisi del "Libro verde sulla spesa pubblica". La politica del centro-sinistra è faziosa e velleitaria, signor Presidente, perché fin dal primo giorno ha perseguito fini di parte e di potere prima che gli interessi generali. Il no dell'UDC alla Nota di aggiornamento è pertanto un no di merito, per le la ragioni dette, ma anche un no politico, per il giudizio negativo che gli italiani - otto su dieci - danno prima di noi sulla cattiva politica di questo centro-sinistra.

richiamata dallo stesso Governo nel DPEF medesimo, di fissare una precisa scansione nella riduzione della spesa primaria corrente nei prossimi anni fino al 2011. Il Governo si impegnò in Parlamento a presentare questa scansione, che trovo contenuta nella Tavola 3 della Nota di aggiornamento; quindi, dal punto di vista del rispetto dell'impegno formale, per quanto mi riguarda, ci siamo. Tuttavia, proprio da quella scansione della spesa primaria corrente che emerge nella Tavola 3 credo dobbiamo riconoscere che emergono elementi di preoccupazione. Ciò vuol dire - abbiamo ascoltato anche ieri il ministro

un obiettivo di pareggio di bilancio per il termine di questa legislatura, per il 2011. È opportuno che così avvenga, e così fa la Nota di aggiornamento. Dobbiamo riconoscere che questo obiettivo non può essere raggiunto con un innalzamento della pressione fiscale, che ha già raggiunto livelli molto alti nel nostro Paese. Dobbiamo aggiungere che non è assolutamente proponibile immaginare di raggiungerlo attraverso una riduzione della spesa per investimenti. Il Ministro dell'economia ha già ricordato che

Il livello dei tassi di interesse, ovviamente, è determinato dal mercato, il livello della spesa per interessi è determinato dal mercato e dal livello del debito, l'unica variabile da utilizzare per raggiungere il pareggio di bilancio è costituito dalla riduzione della spesa primaria corrente. Ora, quello che risulta dalla Tavola 3, purtroppo, è che, mentre se fossimo partiti dal 2007 per raggiungere l'obiettivo di pareggio del bilancio agendo sulla spesa primaria corrente avremmo dovuto ridurre, se i miei conti sono giusti, di 2,7 punti percentuali di PIL la spesa da

Qual è il punto? Abbiamo meno tempo per fare un percorso, che addirittura è un po' più lungo, di riduzione della spesa primaria corrente. Nei conti che il Governo ci presenta per raggiungere l'obiettivo di pareggio di bilancio con quei vincoli sarà necessario ridurre di 2,8 punti la spesa primaria corrente in tre anni. Chiunque abbia maneggiato la finanza pubblica si rende conto di quanto questo impegno sia gravoso,

di revisione radicale dei confini e della dimensione dell'intervento pubblico in economia e di ridefinizione dei meccanismi attraverso cui esso viene realizzato. Me lo conferma il fatto che gli unici anni recenti in cui, in effetti, il livello della spesa primaria corrente in rapporto al prodotto si è ridotto in modo consistente sono gli anni 1993-1995, anni nei quali fu compiuta una vasta opera di ridimensionamento dell'intervento pubblico in economia e furono riformati alla radice alcuni meccanismi attraverso cui questo intervento si compie. compie. Ho ascoltato anche il Ministro dell'economia osservare che non tutto può essere fatto in finanziaria. Credo sia così, anzi, sempre meno dovremo cercare di fare in finanziaria.

Credo sarebbe opportuno, ad esempio, che il Parlamento impegnasse il Governo a riferire ogni tre mesi sullo stadio al quale sono giunte le sue elaborazioni e le sue proposte, con riferimento alla necessità, che il Governo stesso dichiara, di ridurre di quasi tre punti in tre anni la spesa pubblica in rapporto all'economia. Concludendo, vorrei rivolgere una specifica domanda al Governo, alla cortesia del sottosegretario Sartor. Registro nella relazione previsionale e programmatica un andamento del deflatore del Prodotto interno lordo di circa il 2,4, se ben ricordo. di una differenza abbastanza consistente rispetto al deflatore dei consumi o comunque degli impieghi interni delle risorse. Mi chiedo se quel numero non sia eccessivo, considerando anche che sostanzialmente l'altezza sostanzialmente l'altezza relativa rispetto all'impiego interno delle risorse è determinata dall'andamento dei prezzi all'esportazione. A me pare difficile che continui ad avvenire nei prossimi anni quanto è accaduto negli anni passati,

che ha colpito - anche dal punto di vista immaginifico - l'America e l'Europa, sostanzialmente si confermano tutti gli obiettivi di finanza pubblica. La Nota e l'intervento ieri del ministro Padoa-Schioppa spiegano bene il perché. Un numero sintetizza tutto: nonostante la manovra espansiva di luglio, il decreto-legge n. 81 del 2007, la Nota migliora il saldo portandolo da meno 2,5 punti di PIL a meno 2,4. In questo senso questo è il secondo aspetto che politicamente vogliamo mettere in evidenza - vengono confermati sostanzialmente tutti gli obiettivi che riguardano la risoluzione del DPEF di luglio. Stante così la situazione, rimandando alla dichiarazione di voto qualche ulteriore considerazione, mi permetto di evidenziare un elemento. Vi è una polemica, che in parte è stata espressa dal collega Baldassarri nella pregiudiziale e in parte ha vissuto nell'intervento del del tutto evidente che la scelta del decreto collegato alla finanziaria, come collegato sostanzialmente tecnico, fa ricadere tutti gli effetti finanziari nel 2007. Questo mi sembra un fatto molto importante. Allo stesso tempo, ho molto apprezzato la riflessione di ieri del Ministro, quando egli

Signor Presidente, forse perché è poco tempo che sono in Senato, riesco ancora qualche volta a stupirmi. Ieri, mi sono stupito per la qualità e la durata dell'applauso che la mia parte ha dedicato al ministro Padoa-Schioppa. Ci siamo resi conto, credo, che abbiamo alla guida dell'economia italiana un buon pilota, che sa dove andare, per quali strade, in quali tempi, senza scossoni,

quali notizie, quali novità contiene questa Nota. Non sono notizie la crisi dei mutui *subprime* e il rallentamento della crescita del PIL 2007-2008 che si prevede ne consegua. Non sono notizie il miglioramento dei conti pubblici, già anticipato in sede di legge di assestamento, e in particolare nell'ultimo emendamento governativo. Forse non è neppure notizia, in senso proprio, l'utilizzo che nel 2007 viene fatto dei soldi che si pensa ci siano in più: abbassamento del *deficit* previsto dal 2,5 al 2,4 per cento, investimenti in infrastrutture, aiuti agli incapienti, impegni internazionali, anticipo del rinnovo contrattuale. Si tratta di utilizzi del tutto coerenti con gli obiettivi del Governo (risanamento, sviluppo, equità) e, soprattutto, come ha ricordato il senatore Tecce, con il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per Sul piano politico, certo, è possibile dissentire da queste scelte o rammaricarsi che l'enfasi su ciascuna delle tre direttrici avrebbe potuto essere diversa. Non si può però accusare il Governo di incoerenza.

con una curva più lineare, meno tendente verso la fine del periodo, rispetto a quella disegnata dal DPEF. La terza novità è che la spesa pubblica primaria migliora in qualità. Secondo il DPEF, nel 2007 si prospettava una spesa in conto capitale del 9,49 per cento delle spese totali, al di fuori degli interessi.

10 miliardi dei debiti pregressi, precedenti al 2005, delle Regioni vengono ristrutturati e ricontrattati a tasso migliore, con l'intervento dello Stato. È un'operazione conveniente per il sistema finanziario della pubblica amministrazione, che consente di fare chiarezza nei conti regionali. Si tratta anche di un'operazione di moralizzazione, se hanno fondamento le recenti inchieste giornalistiche sulle cartolarizzazioni di alcune Regioni. Nonostante le apparenze, è un'operazione indispensabile per far passare il federalismo fiscale da formula retorica a prassi amministrativa.

finanziaria e del precedente Documento di programmazione economico-finanziaria di questo Governo? Il ministro Padoa-Schioppa si presenta l'anno scorso al Parlamento, dicendo che la situazione è assolutamente avviata verso il disastro, che in tutti i decenni passati nulla è stato fatto e che la nostra stella polare dev'essere la metodica di conduzione della politica economica

della ricchezza e come allocazione di risorse per migliorare la produzione e lo sviluppo non avevano sortito risultati, l'unico metodo possibile e innovativo era quello della riduzione del debito pubblico.

presentata una finanziaria pesantissima, da 35 miliardi di euro. Dunque, il ministro Padoa-Schioppa vuole presentarsi allo scenario nazionale e internazionale, con la sua storia di *commis* economico italiano ed europeo, come un novello risanatore della finanza pubblica, come un novello Marco Minghetti, se non fosse che molti storici hanno dubbi sulla qualificazione e sulle qualità di quest'ultimo, perché sembrerebbe che abbia risolto i problemi dell'allora novella Nazione italiana risanando i conti pubblici con il tesoro del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. E allora, cosa fa il ministro Padoa-Schioppa? il ministro Padoa-Schioppa? Comincia a mettere le mani nelle tasche degli italiani, con un'azione di aumento della pressione fiscale incredibile ed inusitata, portandola ai massimi storici. alla prima bugia: «Le cose vanno malissimo», aggiunge una seconda bugia: «Non aumenteremo le tasse». La prima bugia è risultata evidente perché

caratteristiche ed anche la consistenza, vista la difficoltà del Governo nel produrre i dati che hanno realizzato la proposta di una nuova sistematica al bilancio dello Stato attraverso l'assestamento, l'Esecutivo ha utilizzato queste risorse. Bene fa

questo eufemismo in politica equivale a dire che si sono fatti regalie e sperperi. La redistribuzione sociale, infatti, nell'utilizzazione delle risorse di cui al predetto decreto, non ha significato un uso delle risorse per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta, ma ha significato rimediare ad errori compiuti nella stesura del bilancio precedente, facendo quindi tornare ai Comuni quanto era stato

si coprono questi 18,5 miliardi? In gran parte, per più di 6 miliardi di euro, con risparmi di spesa. Ma se il Governo non è stato capace non è stato capace di mantenere quei risparmi che erano stati quotati nella finanziaria precedente (tanto che, dopo aver accantonato, ha dovuto disaccantonare) come ci può prospettare la possibilità che la finanziaria prossima sia coperta e che quindi il Documento di programmazione economico‑finanziaria individui 6 miliardi di spese come possibile copertura? Ma ci sono tantissime altre cose che non vanno. Ad esempio, il fatto che si vogliano anticipare le spese delle Regioni, trasferendo alle stesse, come anticipazione di cassa, 9 miliardi di euro. Ebbene, signor Presidente, tutti sappiamo che nell'economia banale, anche di tipo familiare, anticipare le uscite significa aumentare le spese e quindi, a questo punto, ci saranno 9 miliardi che peseranno sulla cassa: 9 miliardi che vanno a pesare sulla cassa significano un aumento del debito pubblico, quindi del carico degli interessi e comportano quindi l'impossibilità di rispettare gli obiettivi di macroeconomia che il Governo si pone. Qual è, allora, la buona sostanza dei fatti? Quella di una finanziaria che viene costruita - di cui parleremo a seguire nei prossimi giorni - con delle individuazioni di grandezze macroeconomiche assolutamente difficili. Il senatore Vegas non vuole che io dica una cosa del genere, ma la verità, signor Presidente, è che, viste le grandi difficoltà a discernere tra i numeri, penso al fatto che per tanto tempo si è detto che, se le cose erano andate meglio di quanto previsto, ciò era da attribuire al famoso "fattore C" del Governo Prodi, cioè a quella parte che non sta né alla testa né ai piedi. Signor Presidente, credo non si tratti del "fattore C" del Governo Prodi, ma alla luce di come stiamo esaminando la finanziaria di un altro "fattore C": quello che - per intenderci con chi ha non ha una merliniana memoria - è riferibile ad una casa un po' più piccola con la "o" finale. Signor Presidente, la Nota di aggiornamento dimostra alcune cose e in particolare modo quanto ha sostenuto negli ultimi mesi il senatore Baldassarri sul fatto che nel bilancio dello Stato siano state sottostimate le entrate. Basta fare un paragone tra il Documento di programmazione economico-finanziaria originario approvato e questa Nota di aggiornamento:

Ecco, quindi, che il grande can-can sul recupero dell'evasione fiscale altro non è che una iniziale sottostima delle entrate, attualmente verificate su importi maggiori: è una politica di bilancio volta a nascondere e ad evitare, per quanto era stato enunciato all'inizio della legislatura e nella finanziaria scorsa, manovre di correzione, che in questo modo hanno un altro nome, in quanto si riferiscono all'impiego dei cosiddetti tesoretti, su cui viene speso, in maniera assolutamente sbagliata, il recupero dell'evasione fiscale. Nella realtà dei fatti, invece, si tratta di una ridotta valutazione delle entrate originariamente previste. Un'altra osservazione è sull'indebitamento netto. Lasciando perdere il 2006 al 4,4 per cento, dovuto - come sappiamo - anche ad eventi eccezionali in ordine alla finanza pubblica, vediamo che per il 2007 si passa dall'1,9 al -2,4 secondo il tendenziale post decreto‑legge che sta arrivando adesso in Senato.

maggiori entrate che deriva la copertura delle maggiori spese, tant'è che anche nel dato delle imposte dirette 2007 post decreto-legge vi è, rispetto al dato pre decreto‑legge, una diminuzione della previsione delle imposte dirette in entrata dovuta ad una maggiore riduzione fiscale rispetto all'aumento dell'indebitamento netto, così come dimostrato da questi numeri.

da fare capire che la politica di bilancio ha un'ottica assolutamente ristretta. Infatti, non dà dati attendibili per il medio periodo e non fa altro che confermare, sia sotto il profilo della politica delle entrate - quindi la maggiore tassazione - sia dell'aumento delle spese,

ha chiesto alcune delucidazioni e alcuni chiarimenti. Ha chiesto che l'Esecutivo spiegasse alcune cifre e alcuni dati dai quali dipende la credibilità della Nota di variazione al Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'ennesima volta questo Governo non fornisce risposte, rende monco il dibattito politico e non crea, quindi, le condizioni per un rapporto corretto tra maggioranza e opposizione.

e - aggiungo - dell'analisi compiuta e puntuale sulla situazione reale che caratterizza oggi il nostro Paese. In riferimento, invece, alla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria

come sia improvvisata la vostra politica economica. Il secondo: questo Governo non ha una strategia in tema di riduzione del debito pubblico, che è uno dei grandi problemi e dei grandi macigni che gravano sul nostro Paese. Il terzo: la tendenza a trasferire nel tempo le grandi questioni che affliggono l'Italia. Ma questa è materia di dibattito politico e sarebbe troppo facile per me e per l'opposizione dire in maniera molto chiara che la tendenza a questa propensione propensione nasce dalla consapevolezza delle divisioni e delle lacerazioni che oggi caratterizzano la maggioranza. Divisioni e lacerazioni che solo in alcuni momenti vengono sopite, ma che, di fatto, stanno facendo arretrare il nostro Paese. Quest'ultimo, invece, dovrebbe cogliere, soprattutto in momenti particolari come questo, l'occasione per far compiere un salto di qualità alla propria programmazione e al proprio futuro.

Una differenza dello 0,4 per cento che si traduce in circa il 20 per cento della crescita complessiva di quest'anno e che, quindi, verrà meno l'anno a venire. Ciò a dimostrazione che non state adottando una politica virtuosa e che questo Paese arretrerà sempre di più. cento che conferma quanto sia sciagurata la vostra impostazione tecnica ed economica, che non è possibile superare come fattore, nonostante il Ministro dell'economia, che assume ormai ogni giorno di più i panni del provocatore, così come ha fatto ieri nel corso del suo intervento qui in Senato, sia ormai solamente propenso e disponibile alla "politica del torcicollo", cioè a guardare solamente al passato e a cercare di scaricare sul passato responsabilità che, invece, sono di questo Governo e di questa maggioranza. Emerge, quindi, dalla Nota di aggiornamento la miopia del vostro progetto politico. Devo dire che non ne siamo meravigliati perché non avete affrontato in maniera puntuale e analitica alcune questioni che, comunque, sono sotto gli occhi della pubblica opinione e dei più accorsati osservatori di cose politiche e di cose economiche.

Si è creato ed agitato il fantasma e lo spauracchio del 1929. Nessuno però ha detto in maniera specifica se questo disastro di natura

senza entrare nel merito, senza sfaccettarlo e segmentarlo come sarebbe stato opportuno, così come siete abituati a fare in un processo di approssimazione dell'analisi e quindi anche delle sintesi politiche ed economiche. Non è stato affrontato in maniera analitica neanche il problema dell'apprezzamento dell'euro: è vero che, sotto certi aspetti, esso ci espone in maniera negativa sul piano delle esportazioni, ma è vero di converso che in alcune circostanze può creare un volano virtuoso per la crescita della nostra economia e per l'apprezzamento del nostro sistema Paese.

Se voi aveste pensato soltanto per un attimo in maniera molto seria ad una vera programmazione del sistema economico del Paese, non avreste dovuto trascurare

al contrario, di fatto hanno dimostrato quanto noi stiamo ripetendo da molto tempo, cioè che l'extragettito, soprattutto quello derivante

di fare emergere tutte le falsità e le mistificazioni che si stanno determinando negli ultimi tempi. Ad esempio, quando la modestissima riduzione dell'IRES è più che compensata dall'ampliamento della base imponibile, non si può affermare di avere svolto un'azione virtuosa a favore delle imprese; quando gli interventi sull'ICI vengono più che compensati dall'incremento delle rendite catastali (con i catasti ormai passati ai Comuni), si deve dire tutta la verità fino in fondo e per intero, evidenziando che sugli enti locali

ma di fronte all'ennesimo goffo tentativo di celare le debolezze di questo Governo e di questa maggioranza.

Tuttavia, signor Presidente, insisto su un altro dato. Con la finanziaria che esamineremo nei prossimi giorni la pressione fiscale per l'anno prossimo viene stabilizzata e l'obiettivo del Governo e di questa maggioranza, quale emerge

un dato e dire che l'aumento della pressione fiscale derivi dal fatto che, a parità di aliquote, chi già pagava adesso paga di più perché non è vero.

La seconda questione riguarda il fatto che il tendenziale del *deficit*, come avevo già tentato di illustrare nella relazione,

alle future generazioni e per questo dobbiamo ridurlo. Inoltre, c'è la questione della competitività nei confronti dei nostri *partners*. Se noi spendiamo 70 miliardi di

Circa il dibattito che si è svolto in Aula, desidero anch'io fornire alcuni elementi di replica, partendo dagli aspetti giù generali e soprattutto ricordando qual era il quadro di finanza pubblica che si è andato delineando negli ultimi anni, prima che l'attuale Esecutivo Va ricordato, innanzi tutto, che la spesa corrente era completamente fuori controllo e i tassi di crescita che sono riportati nei documenti lo testimoniano; si è verificata una riduzione della spesa per infrastrutture nonostante i programmi nominalistici che ne prevedevano l'espansione; il debito pubblico ha aumentato la propria incidenza sul PIL, invertendo quindi quel percorso di rientro che era stato avviato già all'inizio degli anni Novanta, e soprattutto esisteva una diffusa sensazione di impunità tra gli evasori, giustificata da un ampio e persistente ricorso ai condoni. Ora questa tendenza è stata invertita in termini e in tempi estremamente rapidi e con azioni significative. Per tutti valga osservare la situazione che caratterizza la spesa sanitaria: con la firma del patto per la salute, che ha stipulato un accordo e un impegno tra Governo e Regioni, la spesa è stata posta sotto controllo e ridurrà la propria incidenza sul PIL mantenendo appena crescente la spesa in valore assoluto. un'inversione di tendenza radicale rispetto a quanto osservato negli anni precedenti. Non solo, ma le operazioni finanziarie straordinarie che sono state già in parte poste in essere questa primavera e che si proporranno con decreto e con il disegno di legge finanziaria sottolineano la situazione di profondo squilibrio finanziario che si era andata recando negli anni successivi, costringendo addirittura il Governo a proporre forme di ristrutturazione del debito che altrimenti si rivelerebbero insostenibili per le Regioni. Questa è la situazione dei conti di finanza pubblica che si era andata delineando e che è stata rapidamente invertita. Per quanto riguarda il Documento che è ora all'esame dell'Aula, va sottolineato il miglioramento dei saldi rispetto agli obiettivi concordati dalla Comunità Europea, nonostante vi sia una crescita economica meno favorevole del previsto; quindi, una parte del miglioramento dei conti pubblici è anche destinata alla riduzione del *deficit* di un punto decimale. A questo proposito, anche per fare chiarezza sulle questioni relative agli effetti di manovre *una tantum* del passato, vanno citati due dati riportati nelle tabelle del Documento. Il primo è che l'indebitamento netto, al netto delle *una tantum* e degli effetti ciclici, quindi calcolato secondo le metodologie standardizzate della Comunità Europea, era pari al 2,8 per cento nel 2006, sarà pari al 2,3 per cento per cento nel 2008. Quindi, depurato dagli effetti della crescita economica e dagli effetti dei provvedimenti *una tantum*, vi è un sostanzialmente miglioramento dei conti pubblici. Lo stesso si può dire, ed anzi in termini quantitativi è ancora più forte, se si osserva l'avanzo primario corretto per il ciclo. L'avanzo primario era di solo 0,6 punti percentuali del PIL nel 2006, è stato riportato al 2,7 per cento nel 2007 e sarà pari al 2,9 per cento sono i segni concreti e tangibili dell'azione di risanamento dei conti pubblici. Ma ancora più importante è il processo di riqualificazione della spesa a favore delle infrastrutture materiali ed immateriali. Dobbiamo ricordare la manovra d'urgenza che è stata fatta nella primavera del 2006 proprio per evitare che si bloccassero bloccassero i cantieri aperti per la viabilità stradale e ferroviaria in seguito alla carenza dei fondi. Una volta ripristinata la situazione di normalità con l'utilizzo in parte delle maggiori risorse, proprio per prudenza, non avendo ancora certezza circa il grado di continuità di queste risorse, si proporrà al Parlamento una serie di opere infrastrutturali, sia a livello nazionale sia a livello locale, contribuendo anche per questa via alla crescita dell'economia. Fatte queste premesse di tipo generale penso di potermi soffermare su alcuni chiarimenti chiesti nei vari interventi.

attraverso l'emendamento all'assestamento di bilancio e attraverso la presentazione di questi documenti c'è un allineamento perfetto tra le previsioni di entrate tributarie e contributive del bilancio dello Stato e i documenti di politica economica. Circa la presunta irregolarità nella copertura dei provvedimenti d'urgenza proposti,

desidero ricordare - anzitutto a me stesso - la distinzione tra accertamento di maggiori entrate e assestamento. L'accertamento di maggiori entrate è un atto obbligatorio, che altrimenti potrebbe portare ad un reato di grave danno erariale ed è sufficiente a consentire l'utilizzo delle stesse entrate mediante disposizioni di legge. Questo è l'accertamento; diverso è il caso dell'assestamento, che è un atto discrezionale con cui il Governo può aggiornare le previsioni di bilancio in corso d'anno. per trasparenza e per rispetto del Parlamento, il Governo ha deciso di assestare il bilancio al fine di allineare le previsioni contenute nel bilancio con quanto è già stato accertato, in quanto effettivamente introitato. Quindi, con assoluta fermezza va respinta ogni possibile ipotesi di irregolarità nelle forme di copertura dei provvedimenti posti all'attenzione del Parlamento. Infine, un accenno alla questione sollevata dal senatore D'Amico circa le previsioni macroeconomiche. Desidero precisare che le previsioni macroeconomiche non sono frutto di un'analisi compiuta esclusivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma rappresentano un atto di consenso che coinvolge i principali istituti di analisi pubblici e privati. L'andamento del deflatore delle esportazioni, più dinamico rispetto a quello dei consumi interni, fondamentalmente riflette riflette il processo di riqualificazione della produzione dell'industria italiana nei confronti dell'estero, giustificato da un desiderio di collocarsi in segmenti di mercato più remunerativi. Quindi, questa divergenza riflette delle

Abbiamo concluso il dibattito;

all'articolo 1, comma 4, alla presentazione della relazione sul gettito tributario e, in particolare, sull'andamento delle entrate rispetto all'evasione fiscale, per dare per dare al Parlamento cognizioni sulla dinamica dell'aspetto strutturale rispetto a ciò che proveniva dalla lotta all'evasione. Il senatore Ripamonti, nella sua replica, ha auspicato che questo Documento sia presentato nei prossimi giorni. Chiedo, pertanto, Presidente, il suo intervento affinché il Governo presenti al più presto

dell'extragettito, la natura della parte strutturale e quella, invece, relativa al CICR, è stata chiesta al Governo in Commissione bilancio. Il vice ministro Visco si è impegnato a presentarla nei prossimi giorni.

conoscendo il suo zelo e il suo rigore nella conduzione dei lavori, vorrei rammentarle che se il rappresentante del Gruppo che deve fare la dichiarazione di voto è assente, decade. Siccome siamo abituati, in questa Aula, ad un atteggiamento

la seduta è ripresa. Colleghi, sono scaduti i tempi per la consegna degli emendamenti.

Presidente, direi che la pausa che lei ha annunciato ben si intona con quanto sto per dire. Vorrei rivelare dove si trova in questo momento il presidente del Senato Marini. è sul Colle di Miravalle, a Rovereto, in Trentino, dove è ospite d'onore di una cerimonia davvero significativa. Oggi ricorre l'ottantaduesimo anniversario del primo rintocco di Maria Dolens, che - per chi non lo sapesse è la campana più grande del mondo che suoni a distesa. Fu ricavata con la fusione dei cannoni dei Paesi belligeranti nella Prima guerra mondiale e ogni sera, alle ore 18, dal colle che sovrasta la città di Rovereto, manda cento rintocchi in tutte le valli del Trentino e, quando il vento è favorevole, fino nelle limitrofe vallate del Veneto. In questo momento, si sta svolgendo una grandissima cerimonia, con la partecipazione

partecipasse idealmente, anche se da lontano, a questo momento particolarmente significativo, che ricorda i motivi di pace che Maria Dolens ogni sera richiama con i suoi rintocchi. *(Applausi

poco fa. È deceduto l'agente del SISMI Lorenzo D'Auria, che era rimasto gravemente ferito in Afghanistan. A nome di tutti, esprimo il dolore di questa Assemblea e il cordoglio ai familiari e chiedo che

La Presidenza ha già sollecitato il Governo perché possa venire a riferire. Mi auguro che ciò sia possibile, visto che i tempi probabilmente lo consentiranno,

e la finanziaria stessa, nonchè il disegno di legge di assestamento di bilancio (che mi auguro voteremo nei prossimi giorni) costituiscono tre fasi dello stesso processo di costruzione della decisione di bilancio 2008-2010, il saldo netto del bilancio 2008 presuppone che gli interventi recati dal decreto-legge siano effettuati con le modalità previste dallo stesso decreto-legge nel 2007. Ciò costituisce, nell'impostazione della manovra, una precondizione tecnico-operativa per chiudere i saldi 2008-2010 all'interno del *target* indicato nell'articolo 1 della legge finanziaria. Per quanto

tale rapporto rispetto alle tabelle previste dalla Nota di aggiornamento, portandolo al 39,3 nel 2008, al 38,7 nel 2009, al 38 nel 2010 e al 37,2 nel 2011,

complessivamente rispetto alle tre questioni che attengono alla linea di politica economica del Governo, cioè risanamento, equità e sviluppo, ritiene corretti

ritengo l'emendamento non ammissibile. In ogni caso, ritengo improprio che si possa intervenire con una risoluzione sulla Nota di aggiornamento per indicare cosa

il tema delle indennità spettanti ai membri del Parlamento è già oggetto della finanziaria, credo che l'esame

Signor Presidente, in merito all'emendamento 2.1, se sotto il profilo qualitativo può essere condivisibile l'invito a contenere la spesa primaria corrente, va peraltro sottolineato come i limiti quantitativi inseriti nella Nota di aggiornamento appaiono adeguati alla luce della concreta attuabilità, per cui il parere è contrario. Sull'emendamento 2.2 mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Il tema della dimensione dell'Esecutivo è tipicamente oggetto di dibattito politico e non appare invece adatto ad essere inserito in un quadro programmatico che è tipicamente contenuto nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria e che riguarda principalmente gli aspetti macrofinanziari e macro-economici. Per questi motivi il parere è contrario. esprimo un parere contrario sull'emendamento 2.3, in quanto nel disegno di legge finanziaria è contenuta una precisa proposta del Governo su questi temi ed eventuali modifiche saranno deliberate in seguito al dibattito parlamentare.

nella Nota c'è uno specifico riferimento al collegato che, per la parte non inclusa nel disegno di legge finanziaria, interviene sui costi della politica e sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi, è evidente che il riferimento ad uno strumento definito come collegato è altrettanto concreto; così come la parte relativa a quella già contenuta nella legge finanziaria rispetto all'adeguamento delle indennità parlamentari non è identica a quella che viene proposta, trattandosi in quel caso di una misura sospensiva di cinque anni e invece, nel caso dell'indirizzo dato alla

Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 2.2 perché fortemente riduttivo rispetto alle esigenze che si pongono in tema di riduzione dei costi della politica. Riteniamo che la riduzione dei membri del Governo - che vuol dire ripristino della legge Bassanini - ed altre consistenti misure debbano essere approvate già nella legge finanziaria.

proporre quegli incisivi tagli ai costi della politica, compreso il ritorno alla legge Bassanini per il numero dei Ministri e una drastica riduzione del numero dei Sottosegretari, che intendiamo sottoporre all'esame di quest'Aula la prossima settimana, qualunque cosa decida di fare il Governo.

Il primo degli emendamenti affronta il tema della riduzione dei membri dell'attuale Esecutivo. Si tratta di un tema che ha grandissima rilevanza politica e che - a mio avviso - deve essere affrontato in un contesto nel quale, prima di tutto, è necessario, al fine di sviluppare un'iniziativa incalzante per la riduzione dei costi della politica, che il Governo, che questa azione deve guidare, si metta in grado di non prestarsi in partenza, data la sua composizione e il numero dei suoi membri alla più banale ed elementare delle osservazioni: come fa un Governo che ha un numero così elevato di membri a risultare credibile nel proporre al Paese un ridimensionamento drastico dei costi della politica che riguardano altri organi istituzionali e la pubblica amministrazione nel rapporto con gli organismi politici nel suo nel suo complesso. Indubbiamente, quindi, l'intervento per la riorganizzazione del Governo in una chiave - ripeto - volta a conferirgli la credibilità necessaria per sviluppare un'iniziativa di riduzione dei costi della politica,

Presidente) che sostengono che in questo momento la normativa vigente obblighi all'adeguamento automatico delle indennità parlamentari; la mia opinione, invece, è che nella legislazione vigente l'obbligo di adeguamento automatico non esista. Questa è la mia tesi, ma non pretendo che sia condivisa

per i quali per di più si è aggiunto un costo *ad hoc*. Ricordiamo tutti, infatti, che molti senatori, membri del Governo, sono stati invitati a dimettersi da senatori per restare membri di Governo al fine di garantire i numeri in quest'Aula. Ebbene, in quel momento, si è raddoppiato il costo: alcuni lo hanno fatto, altri non lo hanno fatto e sono tuttora membri del Senato e membri del Governo. In quell'istante, il Governo ha raddoppiato il costo caricando il bilancio dello Stato

il Governo ha aumentato arbitrariamente, per garantire a se stesso i risicati numeri del Senato, i costi della politica.

Infatti non mi sembra una gran bella cosa ridurre, in finanziaria, per contenere i costi della politica, le Assemblee elettive di Comuni ed Enti locali e ridimensionare i Governi degli Enti locali quando poi chi fa questo non fa un passo indietro nemmeno nelle intenzioni.

se siete veramente d'accordo a ridurre i costi della politica, dando l'esempio e partendo proprio da chi formula queste proposte, cioè dal Governo, da questa maggioranza che ha inteso, in qualche modo, interloquire con l'antipolitica delle piazze che si ritrova intorno a Grillo, per dare risposte concrete e non soltanto per poter fare salotto televisivo e tavole rotonde inutili. È necessario essere credibili verso questo Paese ed è necessario che lo siate per l'intera classe dirigente, per l'intero ceto politico, voi che state al Governo, perché noi dall'opposizione non possiamo che stimolarvi, incalzarvi, ma poi, in concreto, chi ha i numeri per cambiare le regole del gioco, purtroppo, siete voi e voi dovete rispondere all'antipolitica prima di tutti quanti noi. Invece, quando vi si offre un'opportunità, fate finta di niente, fate passi indietro. Questo non è accettabile moralmente prima che politicamente. La vostra credibilità, in questo momento, la state mettendo in discussione prima di tutto voi che l'opposizione, quindi vi facciamo un invito a dire almeno parole precise su questa formulazione.

Mi consentirà, Presidente, di esprimere anche un'opinione su quello che ho ascoltato da parte dei Gruppi del centro-sinistra. Qui bisogna ascoltarsi e non dileggiarsi, presidente Formisano e presidente Salvi. Vedete, voi che avete l'opportunità di andare spesso in televisione

che prendete le distanze dai costi della politica. Lo fa il senatore Salvi, che ad ogni finanziaria presenta emendamenti, annunciando i «*penultimatum*» al Governo e adesso avete scoperto questo giochetto anche voi dell'Italia dei Valori. Allora io vorrei sapere di quali valori si sta parlando: se è un valore la bugia di fronte ai cittadini ogni volta che c'è una telecamera della RAI, se è un valore la fuga rispetto alle responsabilità che avete, perché bisognerà pur far arrivare il momento in cui alla parola data corrisponde il fatto avvenuto; con voi non accade mai. *(Applausi del se è vero quello che abbiamo ascoltato ieri, senatore Formisano, dal suo Ministro, perché il suo Ministro ha parlato nel corso della conferenza stampa cui ha fatto riferimento lei, con un atteggiamento poco garbato nei confronti dell'onorevole Fini, e non mi crea problemi il fatto di doverlo difendere rispetto ad un'accusa insulsa che lei potrebbe risparmiarsi.

detto che bisogna ridurre Ministri e Sottosegretari, ha detto che il suo Ministero è a disposizione, che sono a disposizione almeno due Sottosegretari (non so quanti ne abbiate nella spartizione dei 103), e adesso, in Aula, lei fugge e nega quello che ha detto il suo Ministro? Ma in che mondo vivete?

Se vuole essere coerente, almeno si astenga dal partecipare al voto. Faccia come fanno i senatori a vita, che oggi avete dimenticato di precettare per salvare questo Governo che non sta in piedi. Faccia il suo dovere, sia coerente con le parole che ha pronunciato in televisione, perché altrimenti non sarete più credibili. Voglio dire, infine, Presidente, che tra i costi della politica - e penso di aver illustrato le motivazioni per cui siamo con convinzione a favore della proposta sono anche degli abusi che inquietano i cittadini. Spero sia data presto risposta ad un'interrogazione che ho presentato oggi e che riguarda il ministro Mastella.

In quest'Aula si è fatto un processo contro il senatore Selva e occorre allora che il ministro Mastella ci dica se la trasmissione televisiva di Bruno Vespa è più importante del Senato. È inaccettabile che ci sia tale abuso da parte delle cariche di Governo e credo che qualcuno oggi debba fare una riflessione in proposito. Vogliamo sapere se almeno in questo caso la solerte procura di Roma aprirà un fascicolo anche nei confronti del suo Ministro preferito.

specificare due concetti. Il primo è che siamo abituati ai cavalli di Troia del senatore Calderoli - non del presidente Calderoli - che, attraverso ordini del giorno o emendamenti, cerca di incunearsi nelle fila nemiche per gettare scompiglio. la prima motivazione per cui non posso votare a favore e non posso nemmeno ragionare su una non partecipazione al voto è che in qualche modo avallerei un atteggiamento non molto leale.

e si preferisce ragionare su una riduzione del numero dei parlamentari, obbiettivamente, in qualche modo si sfiora il ridicolo. Vogliamo invece che venga recuperata una credibilità complessiva della politica. A questo proposito, abbiamo presentato da tempo

non è necessario fare riferimento al collegato. Capisco che la proposta del senatore Calderoli, in questo caso, non del presidente Calderoli, deve tener conto del contesto nel quale viene formulata: ecco perché c'è il riferimento alla risoluzione e quindi al collegato; però, riteniamo che invece questo sia uno dei temi sui quali concretamente sarà possibile, anche nel contesto della finanziaria, misurarsi in Aula. E quello sarà

il Governo ha provveduto a tagliare le spese di moltissimi Ministeri con un taglio orizzontale, che molto spesso penalizza ambiti e settori che non dovrebbero esserlo, questo stesso taglio orizzontale - lo abbiamo chiesto formalmente al Presidente del Consiglio - noi vorremmo che venisse applicato al Governo. Queste sono le motivazioni che mi inducono a dire che accetteremo la sfida per la finanziaria. Si vedrà in quel contesto chi avrà la forza e il coraggio di sostenere le parole con comportamenti concludenti.

il collega Calderoli spesso presenta delle trappole, però, le garantisco che mi ha detto che stavolta pensava che l'emendamento lo votassero proprio tutti e che non voleva dividere alcunché.

Presidente, innanzitutto vorrei dire al senatore Formisano che noi apparteniamo ad una storia e ad una vicenda politica che ha sempre avuto un rapporto con l'impegno politico in termini di rigore, di sobrietà e di politica intesa come servizio. Non dovevamo attendere il senatore Di Pietro per scoprire il tema del costo della politica e la contestazione e degenerazione dello Stato lottizzato e "clientelizzato" dal Governo di cui fanno parte il senatore di Pietro ed il senatore Formisano. Lo dico per chiarezza perché possiamo anche avere occasionali convergenze, ma non potremo mai avere una strategica convergenza con chi rappresenta un modo di rispondere ad una crisi di sistema cercando di cavalcare con la demagogia e l'ipocrisia e con l'assenza dell'esempio la legittima esigenza di riforma della politica.

la riflessione che a nome del Gruppo sto cercando di rendere con chiarezza al Parlamento, all'alleanza di centro destra, di cui facciamo parte. Ciò detto aggiungo, per estrema chiarezza, senatore Manzione: è un costo della politica fatto anche dell'ipocrisia rispetto alle questioni ed ai problemi. Non è possibile che ogni volta si cerchi di sfuggire al sì e al no, alla presa di posizione. È ipocrita dire che il senatore Calderoli cerchi il cavallo di Troia: il senatore Calderoli fa una provocazione giusta ed il Parlamento farebbe bene ad accompagnare con chiarezza questa provocazione. La verità è che c'è il riflesso condizionato nel centro-sinistra

- lo voglio dire in particolare ai deputati meridionali - a quanto denunciato, oltre un anno fa, dal presidente della Repubblica Napolitano, il quale, alla Fiera del Levante di Bari, inascoltato dal centro-sinistra, che ogni volta utilizza il Presidente della Repubblica, pose una grande questione di sistema, parlando della degenerazione della politica nel Mezzogiorno, nel Mezzogiorno di Bassolino, di Loiero e di Vendola.

sbagliato. Care colleghe e colleghi, credo dovremmo riflettere un momento su questo punto, perché nel rapporto con il Paese siamo chiamati, questo è almeno il mio pieno convincimento, ad operare una svolta profonda nel nostro modo di fare politica, di vivere le istituzioni e di rappresentarle. Non voglio adesso richiamare questioni di principio e di fondo, perché non è questa l'occasione, penso però che dovremmo avere tutti in questa circostanza, o anche in questa circostanza, un po' di prudenza e di cautela. Per esempio, ho trovato un po' singolare - non me ne abbiano i colleghi dell'Italia dei Valori - che un Ministro in carica, che è capo di un movimento politico e di un partito, abbia assunto sul tema dei costi della politica un'iniziativa politica, quindi fuori dal Governo di cui fa parte, fuori del Parlamento di cui è membro, fuori della maggioranza di cui è autorevole protagonista, tesa ad affrontare in termini risolutivi, questo era il suo intento, il tema dei costi della politica, insieme al capo di un altro partito, che però è anche uno dei capi della coalizione

Detto questo, credo sia giusto rivendicare una svolta profonda, nella quale possono essere contenute anche le proposte che il senatore Calderoli ha formulato. Vorrei dire, però, non solo al collega Calderoli, ma anche ad altri colleghi, che se vogliamo affrontare in termini di risposta vera e autentica quella domanda di trasparenza, di rigore, di sobrietà e di austerità che viene nei nostri confronti e più in generale nel modo di essere dello Stato e delle nostre istituzioni, allora e dovrebbe il Governo, magari in occasione della legge finanziaria, presentare un organico piano di proposte che riguardi i costi della politica in senso stretto, che riguardi noi o gli eletti ad ogni consesso, che riguardi i costi delle istituzioni in quanto apparati, in quanto organizzazioni istituzionali. Ad esempio - lo dico per inciso a chi ci ascolta ascolta - i vitalizi o le indennità di cui ci gioviamo incidono nel bilancio del Senato soltanto per il 12 ai costi delle istituzioni, di tutte le istituzioni del nostro Paese e, allo stesso tempo, ai costi della democrazia, che va sostenuta - badate - con la spesa pubblica, così come devono essere efficienti le istituzioni, come dev'essere trasparente la politica. *(Applausi dal

sollecitando il Governo a presentare un piano e un programma di riduzione della spesa che riguarda i costi della politica, i costi delle istituzioni e i costi della democrazia. In tal modo, non dico tutti, ma coloro che hanno la responsabilità di essere classe dirigente a diversi livelli di questo Paese darebbero un contributo di trasparenza e di austerità, che ci viene chiesto in questo momento. Per queste ragioni, non posso votare quell'emendamento che è stato proposto, non per ciò che c'è, per certi versi, ma per ciò che al contrario non c'è.

Pietro. In fondo - lo dico ai miei colleghi Ciccanti e Storace - non bisogna essere così cattivi. Ieri è accaduta una cosa importante, che i *mass media* non hanno rilevato

e come hanno declamato ieri nelle loro motivazioni i suoi amici, la loro intenzione, con l'astensione, era

equivale a un voto contro, contro la nostra richiesta di stigmatizzare e diminuire le spese. Loro non volevano né non stigmatizzare, né non diminuire le spese: volevano fare una cosa diversa da quella del Governo che sostengono.

Anche di questo prendiamo atto: sorge una protesta, non qualunquista come quella del comico, ma seria nel cuore e nella testa dei parlamentari contro il Governo che sostengono. Questo sta accadendo in più parti della maggioranza, perché è giusto, in effetti, agire subito con l'organo che può farlo, cioè il Governo, verso un'esigenza che tutti sentono. Il ministro Santagata è stato il più comico di tutti,

due i motivi: probabilmente allungarsi la vita; in secondo luogo, andare incontro alla richiesta populista di Grillo, in un modo ancora più populista.

Deve concludere, senatore Sono arrivati un po' tardi, però l'importante è che abbiano rilevato che il nostro contributo, anche secondo loro, è utile.

prevede una riduzione dei costi della politica per non meno di 2 miliardi. È un'iniziativa che soprattutto questa parte politica ha proprio perché il tema non poteva essere rinviato. Condivido quindi quanto ha affermato prima il senatore Salvi. Noi siamo contrari su questo emendamento, anche nel testo riformulato dal collega Polledri, perché vogliamo che ci sia un intervento globale di non meno di 2 miliardi di risparmio. Quindi, evitiamo improvvisazioni o strumentalizzazioni:

si salvaguarda la funzione propria di questa Nota di aggiornamento, che è quella di informarci sulle novità intervenute sull'indebitamento netto (che è diminuito di un decimo di punto, ma sembra che nessuno se ne occupi) e sulle previsioni di crescita, e si fa chiarezza.

delle Comunità montane e delle Regioni meridionali, senatore Viespoli. Al senatore Viespoli però voglio chiedere di non fare facili strumentalizzazioni. Noi non abbiamo esitato a denunciare limiti ed errori gravi anche di alcune Regioni meridionali oggi governate dal centro-sinistra. In quest'Aula, alcuni nostri esponenti hanno attaccato fortemente, ad esempio,

Non certo perché abbandoniamo una battaglia che da almeno due anni abbiamo iniziato, ben prima che giornalisti autorevoli e comici scendessero in politica - lo dico anche senza alcun intento di censura - e ben prima che quest'Aula ne prendesse consapevolezza. Già nell'ultima finanziaria presentammo un nutrito pacchetto di emendamenti che non ebbero una sorte particolarmente felice. Se ci fosse stata allora più attenzione, forse oggi avremmo un comico in più e un politico in meno.

superiore a 50, nel rispetto del principio di genere. Abbiamo dunque una proposta precisa che tradurremo in un emendamento alla legge finanziaria, insieme ad un altro pacchetto di proposte sistematico sui costi della politica. Pensiamo che la finanziaria sia la sede appropriata sia per la riduzione di spesa che questo emendamento produce, sia per la certezza dei tempi che assicura. Quindi confermiamo ai colleghi che hanno manifestato analoghi intendimenti che ci sarà una nostra iniziativa in tal

aumentare i Ministeri, creandone alcuni su misura per alcune forze politiche che hanno sostenuto la sua maggioranza. noi andammo al Governo, Presidente, onorammo la riforma Bassanini, pur costandoci anche in termini di equilibri di coalizione. Ripristinammo solo due Ministeri che si consideravano e sono considerati strategici, quello della salute e quello delle comunicazioni; per il resto la riforma Bassanini è entrata in vigore

Tra l'altro, Presidente, lo spacchettamento selvaggio dei Ministeri, a parte la creazione di Ministeri dei quali nessuno sente il bisogno

di costi. Sui decreti legislativi in merito al riordino dei Ministeri "spacchettati" abbiamo dei pareri dai quali emerge chiaramente che le direzioni e gli uffici di direzione generale dei Ministeri sono aumentati e che la riduzione della passata finanziaria vale solo per i Ministeri così come erano già stati aumentati sulla base dello spacchettamento. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che la finanziaria non sia sede adatta per risolvere questi problemi, ma allora chiedo ai colleghi della maggioranza: è sede adatta la finanziaria a modificare gli organi di Governo delle autonomie locali? quella del Consiglio dei Ministri, ad annunciare, solo per ragioni demagogiche, la riforma costituzionale

Prodi ha dimenticato che tra gli organi costituzionali, come il Parlamento e gli organi periferici, come i consigli comunali,

signor Presidente, cari colleghi, assistiamo ad uno spettacolo che certamente non avvicina l'opinione pubblica al Palazzo o meglio non la avvicina a quella parte dell'emiciclo occupata dal centro-sinistra, perché voi parlate, predicate, dite, annunciate e poi, alla fine, il massimo che fate è astenervi, sapendo benissimo che il voto di astensione - come è stato detto - è un voto contrario e che quindi la vostra maggioranza sarà al riparo da ogni rischio, salvo incidenti di percorso per i quali questo emendamento potrebbe essere approvato. È uno spettacolo veramente indecoroso, del quale noi del centro-destra potremmo anche essere soddisfatti,

le piazze per gli *show* di Grillo, ma tanti cittadini che vorrebbero riconciliarsi con le istituzioni e che vedono invece che in queste Aule si fa tanta, tanta demagogia ma non si producono risultati che possano soddisfare certe esigenze condivise da una grandissima parte del Paese.

che si fanno paladini di certe iniziative e poi, al momento di arrivare al dunque, quando devono dare un segnale concreto, tirano indietro la mano e si scherniscono di fronte ad una situazione che potrebbe mettere in difficoltà il Governo Prodi. Vogliamo accettare la sfida sui costi della politica? Noi siamo pronti a fare il nostro Lo volevamo fare in Commissione affari costituzionali, nella riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. Lo faremo in sede di finanziaria. Ma lo vogliamo fare anche sul punto della riforma della struttura di Governo.

Presidente, ho bisogno di pochissimo tempo, perché ritenevo di dover chiedere pubblicamente scusa ai colleghi senatori di Alleanza Nazionale per l'intervento che ho svolto prima, dove probabilmente le parole hanno tradito il pensiero. Lo faccio, così come ho fatto prima, chiedendo pubblicamente scusa *(Commenti del mi ha colpito l'intensità di alcuni interventi, per cui evidentemente il fatto che le parole abbiano tradito il pensiero ha causato un disagio del quale chiedo scusa in quest'Aula. *(Applausi del senatore solo per dire che non avrei mai immaginato che diventasse centrale la posizione di Italia dei Valori e di Di Pietro: è una constatazione. Rispetto a ciò e a tutte le considerazioni fin qui effettuate, confermo il voto di astensione, non perché non ci sia chiaro che astensione, al Senato, ha una valenza diversa rispetto alla Camera, ma perché le ben note posizioni di Italia dei Valori su questo tema saranno

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, debbo denunciare un profondo malessere in relazione alla discussione che stiamo facendo,

in commistione con la questione degli sprechi, della lotta e dell'economicismo. Rischiamo di far passare l'idea che la democrazia sia un lusso, che la democrazia ha un costo; rischiamo di far passare l'idea che tutto ciò che facciamo e tutto ciò che la democrazia porta

sobria ma non pauperista, sono per razionalizzare il tutto, ma non ci sto che la rappresentanza, le forme di partecipazione delle donne e degli uomini di questo Paese, le forme delle decisioni delegate vengano additate - questo sta succedendo - semplicemente come uno spreco, semplicemente come soldi gettati via, perché questa è la strada maestra che porterà all'idea che allora decide uno

nella nostra umiltà, nei nostri difetti, di rappresentare il benessere di tutta la popolazione, non di quella regione o categoria ma il benessere di tutto il nostro Paese, ma abbiamo anche il dovere di ricordare che su questa strada davvero la democrazia autoritaria e i plebisciti personali sono la via maestra, oltretutto se accompagnati da un sistema integrato delle comunicazioni di massa che ha ridotto il cittadino a semplice utente. Vorrei anche esprimere di fronte a tutti l'orgoglio di essere stato eletto. Non credo di sprecare i soldi, non credo di essere inutile, se lo pensassi mi dimetterei.

il significato di una astensione. Mi astengo perché non esiste alcun altro strumento per esprimere il disagio che si può provare nell'attraversare ancora una volta una mattinata inutile nella quale il Parlamento viene usato come un aereo dirottato e nel quale tutto ciò che era stato stabilito di fare non si è fatto. Leggo, nell'ordine del giorno di oggi:

Ho assistito, invece, ad una serie di discorsi, tipo quelli dell'onorevole del giornalino di Gian Burrasca, che fa appassionatamente il laico e va a sposarsi in chiesa:

Per questa ragione, l'astensione è l'unico strumento con il quale esprimere questo disagio e anche per iniziare a chiedersi se ha senso rappresentare i cittadini

Senatore Colombo, mi permetto di esprimere un'opinione su quello che ha detto. Noi stiamo discutendo un emendamento alla risoluzione alla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria; su questo emendamento vi sono stati interventi assai impegnati e molto seri: penso che possiamo avere tra noi opinioni diverse, ma non credo sia giusto dire che il Senato della Repubblica sta perdendo tempo.

proprio per le questioni ricordate dal senatore Silvestri. Ho sentito stamattina, in un tempo non inutile, sia dal centro‑sinistra sia dal centro‑destra, una maggiore sensibilità al problema dei costi della politica, necessari, come Silvestri ha detto. Probabilmente, però, nel tempo, ci ha preso la mano un vizietto: l'uso del denaro pubblico per il voto di scambio, per le clientele e quant'altro. Se tutti i senatori - e se lo facessero anche i deputati - davvero ragionassero su ciò che avviene dietro le parole e dietro i sacrosanti princìpi che già prima sono stati richiamati, credo che avremmo modo di compiere un passo avanti. Se ricostruiremo un clima in cui io possa liberamente votare l'emendamento della Lega, sarebbe un altro passo avanti.

non vedo santoni all'orizzonte (né Grillo, né Di Pietro). Andrò a cercare un articolo su «La Voce» relativamente a finanziamenti e campagna elettorale trasformatisi in investimenti immobiliari di partiti che annunciano chissà qual rigore (e poi il loro Ministro è quello che ha i maggiori incarichi; abbiamo poi sentito delle Ferrovie dello Stato) né di amministratori che dicono di aver tagliato i consigli di amministrazione (com'è avvenuto in Comune a Ferrara: hanno tagliato due consigli di amministrazione ma poi hanno fatto nascere quattro società composte da tre consiglieri di amministrazione). *(Applausi Concludo dicendo che vi erano tratti del dibattito molto interessanti, ma poi, prima di qua contro Berlusconi, poi di là contro la Campania, siamo tornati avvitarci su questioni di bandiera e di partito.

sull'ordine dei lavori.

"Dopo la parola «Governo», inserire il seguente punto: «a prevedere, già in sede di disegno di legge finanziaria, un ridimensionamento quantitativo dell'Esecutivo e dei relativi costi,

più numeroso, più pesante e più costoso della storia della Repubblica, si contraddirebbe quanto è stato detto tutti i giorni. Oggi lo possiamo fare; se c'è un voto contrario, il Governo sarà autorizzato a non intervenire con il supporto del voto del Senato.

perché ipotizzava che nel collegato, fuori dalla sessione di bilancio, si introducessero norme riguardanti la composizione del Governo in generale.

L'opinione della Presidenza è diversa da quella del senatore Morando. *In primis*, noi stiamo presentando un emendamento alla risoluzione alla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria quindi, non siamo in sede di esame della legge finanziaria. In secondo luogo, dal punto di vista dei possibili riflessi sul piano della spesa e su quello finanziario, è indubbio che la proposta di questo emendamento

del disegno di legge finanziaria, così come presentate dal Governo, presentano questa eccezione di regolamentarità rispetto al riflesso che hanno, o dovrebbero avere,

averlo interrotto contro la mia abitudine - che le origini dello spacchettamento sono nel Governo Berlusconi: con decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, è iniziato lo smantellato della legge Bassanini ed è stato il Governo Berlusconi a superare il numero di 100 membri componenti. Mi fa piacere questo ravvedimento operoso ma ognuno dovrebbe pensare alle cose sue prima di attaccare quelle degli altri.

cioè che sarebbe stato sconveniente procedere ad un automatico aumento delle indennità dei parlamentari, conseguente ad una ad una legge che ha modificato la materia della giustizia. Si dice che nella legge finanziaria è già prevista la sospensione per cinque anni dell'aggiornamento È vero che questo è previsto in sede di finanziaria ma la finanziaria lo sospende per cinque anni mentre la mia richiesta è di intervenire in senso definitivo rispetto a quello che è il tema delle indennità dei parlamentari. Anche perché, non prendiamoci in giro, si è voluto creare un articolo, in risposta forse alle campagne di Grillo, dicendo che questo aumento automatico per cinque anni verrà bloccato. Il problema è che la nostra indennità corrisponde a quella di un magistrato di Cassazione che svolge funzioni dirigenziali. All'interno di questa posizione vi sono 30 gradini e noi siamo collocati a metà. Questo non lo stabilisce la legge ma lo stabiliscono gli Uffici di Presidenza. O si rimette mano, completamente, all'aggancio che noi abbiamo con il Presidente della Corte di cassazione o, viceversa, questa norma manifesto della finanziaria lo bloccherà per cinque anni ma ci sarà tutto lo spazio, negli Uffici di Presidenza, per alzare il livello del gradino e determinare comunque gli stessi effetti senza neppure passare attraverso una legge. Se oggi vogliamo dare un segnale rispetto a quell'aumento, tra l'altro retroattivo, che ci è arrivato - qualcuno diceva addirittura di volerlo devolvere, cosa che tra l'altro è vietata dalla legge credo che si possa dare mandato al Governo, in sede di collegati, di affrontare definitivamente la materia in modo tale che non ci sia la possibilità più per nessuno di nascondersi dietro il dito del fatto che è una cosa che accade per una legge già votata. Quella legge l'avete votata voi, noi abbiamo votato contro quell'aumento di stipendio, cari colleghi.

Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC, sull'emendamento 2.3, indica di votare con libertà di coscienza perché riteniamo che questa sia una prerogativa del Parlamento non delegabile al Governo, facendo un ragionamento che, in qualche modo, vede punti di vista diversi e che dovrà trovare una ulteriore occasione di confronto. Qual è il ragionamento? Il collega Silvestri, nel suo intervento, ha avuto un largo consenso, stando agli applausi ricevuti da tutti gli scranni di quest'Aula, perché ha posto, sul terreno del confronto, una questione: i costi della politica sono diversi dai costi della democrazia e dai costi delle istituzioni democratiche. C'è da una parte uno spreco di risorse dovuto alla duplicazione di uffici derivante da logiche spartitorie:

lei ha giustamente rimbeccato il collega Pastore sul cosiddetto spacchettamento, ma in quell'occasione ricordo che lei insieme ad altri fu fortemente critico sulla revisione della legge Bassanini e anche sul contenuto di merito, sul contenuto politico, di quella decisione presa dal Governo Berlusconi nel 2001.

Tant'è che questa antipolitica è cavalcata soprattutto dalla grande stampa, che è nelle mani dei poteri forti. Non per niente il libro "La casta" è stato scritto da un giornalista che in quell'assetto ha notevoli responsabilità di firma. Tra qualche giorno

che stiamo dando un brutto spettacolo alla pubblica opinione. Non voglio fare demagogia: in Aula non è stato eletto nessuno che risponda al nome di santa Maria Goretti

quale do atto di essere attento perdente su tali questioni, perché non ne vince mai una (ogni volta annuncia battaglia, ma aspetto ancora che risponda su questo tema; fa i "*penultimatum*", ma il Governo resta sempre in piedi, sui costi della politica),

anche questa una logica che non può essere apprezzata dalla pubblica opinione. Ecco perché, senatore Salvi, servono dei segnali. Lei ha detto poc'anzi - e vorrei che glielo ricordassero anche i colleghi che con me sono stati nel Governo Berlusconi - delle inesattezze sul nostro Esecutivo. Ha la compiacenza di ascoltare, magari interrompendo la conversazione con il senatore Brutti, essendo anche una questione di educazione, quando sono poste delle domande? Mi piacerebbe interloquire con il senatore Salvi, ma vedo che non è possibile. Lei ha accusato noi

questo emendamento e vorrei spiegare il perché. Non so chi di voi c'era nel 1992; io c'ero e abbiamo commesso molti errori sull'onda della stessa spinta della piazza che oggi vediamo.

che non si possa derogare dai princìpi fondamentali della democrazia. Uno di questi princìpi è la divisione dei poteri: potere giudiziario, potere esecutivo e potere legislativo, che noi rappresentiamo. Sono assolutamente d'accordo con il contenuto dell'emendamento Calderoli, ma lo ritengo costituzionalmente e tecnicamente sbagliato. Siamo noi, potere legislativo, a dover decidere di noi stessi, altro che delegare il Governo! *(Applausi

il Governo suona le trombe, congelando in finanziaria l'indennità dei parlamentari per cinque anni, e immediatamente l'Aula l'Aula del Senato gli risponde suonando le campane con questo emendamento. C'è uno scavalco verso l'ipocrisia che certamente non fa onore, nemmeno alla classe politica. Mi rendo conto che se qualcuno di noi voterà contro questo emendamento domani sarà attaccato su tutti i giornali, perché, evidentemente, vuole conservare la casta che vuol mantenere ciò che ha ottenuto.

può rincorrere ipocritamente ciò che fuori dalle Aule parlamentari si determina, contro la politica e contro coloro che hanno scelto di fare politica. In quest'Aula, infatti, vi sono senatori che non hanno altre attività, hanno deciso di fare politica da sempre e non possono ascriversi a nessuna casta. Essi hanno

Il senatore Calderoli, che spesso presenta documenti di un certo tipo e che lasciano riflettere, anche in questa circostanza ritengo chieda

voto. Personalmente, voterò contro questo emendamento, con le motivazioni che sono già state esposte dal collega Ciccanti: assistiamo, cioè, ad una replica di quanto alcuni di noi hanno osservato, non da protagonisti, nel 1992 e altri hanno direttamente testimoniato e vissuto. Con l'avvertenza che si tratta di una citazione letteraria, com'è noto, la storia si ripete sempre due volte: la prima in tragedia e la seconda in commedia. Nel 1992 vi fu una tragedia, perché fu travolta una classe politica: cinque partiti furono disciolti attraverso l'azione della magistratura; vi furono suicidi e, in qualche modo, anche omicidi. Una tragedia nazionale di cui paghiamo ancora le conseguenze. Oggi, ad essere benevoli, assistiamo ad una commedia, e non è un caso che a scendere in campo sia un comico che la recita meglio di noi. Io sono stato tra quelli che hanno salutato il suo ingresso in campo con simpatia, ma non c'è nessun bisogno che noi senatori, nell'eccesso di concorrenza, ci mettiamo ad imitarlo. Nella stessa giornata, il Governo dice che i parlamentari per cinque anni cambiano sistema retributivo, il Senato dovrebbe dire "nossignori" per sempre e la Commissione affari costituzionali, stamattina, annuncia che cancella 120 deputati. Signori miei, questa è una sfida al comico Grillo, perché fa ridere che diminuiscano i deputati non avendone i poteri; lo possono fare solo con una legge costituzionale. Credo allora che il rischio non venga dall'antipolitica, da Grillo

nella capacità che non sempre dimostriamo di avere l'orgoglio di svolgere una funzione utile al Paese, con la dignità che ad essa Presidente, darò libertà di voto ai componenti del mio Gruppo, così come ho dato poc'anzi un'indicazione di voto favorevole all'emendamento 2.2 (testo 2), che aveva una sua logica e che, tra l'altro, va in contrapposizione ad un atteggiamento tenuto, paradossalmente, dalla maggioranza, che vota contro una proposta di riduzione dei Ministri e dei Sottosegretari qui in Senato e di contro, alla Camera, vota una proposta che prevede, per il futuro, la riduzione del numero dei parlamentari. riguarda questa proposta, mi sarei atteso, mi attendo e anzi auspico, signor Presidente, un dibattito più ampio, in quest'Aula, sul tema della riduzione dei costi della politica, che deve toccare l'intero sistema pubblico istituzionale del Paese.

sostenendo di doversi ricredere su privilegi che invece in passato sono stati uno strumento di tutela di quel tipo di vita parlamentare che andava assicurato al soggetto che faceva politica, per renderlo impermeabile

senza infingimenti, senza preoccupazioni, ma con l'orgoglio che un potere legislativo deve rimanere immune dai movimenti di piazza, dai movimentismi che non portano da alcuna parte, perché non hanno un progetto di governabilità del Paese.

una risposta politica diretta a bloccare gli automatismi e ad innescare quel meccanismo che, come lei sa, signor Presidente, il Consiglio di Presidenza del Senato ha messo in moto per verificare i costi della democrazia in questo Paese.

Il Senato deve mettersi in condizione non di criticare *a priori* i movimenti che protestano, ma di capire che essi non rappresentano la soluzione e che anche da questi segnali possiamo rigenerare una buona politica, in nome del nostro Paese, che ci chiede questo. È chiaro che i costi della democrazia sono più ampi. È anche chiaro, signor Presidente, che dobbiamo tutelare l'indennità del parlamentare, ma se vogliamo assumere provvedimenti seri, dobbiamo prendere atto

classe politica che mette l'interesse del Paese prima di propri giusti interessi particolari. Devo dire, però, che sarei più contento se il senatore Calderoli lo ritirasse,

oppure non si capisce bene perché i parlamentari vengano considerati particolarmente ricchi in un Paese che morirebbe o affonderebbe.

perché ci obbliga ad un voto discriminato e discriminante, nel senso che, perseguendo lo stesso valore, si possono assumere atteggiamenti che possono apparire contrastanti.

dell'emendamento, ad un gesto che non è un ravvedimemto, ma è la considerazione che un tema come questo debba essere assunto quale programma del Parlamento, per se stesso e per la Nazione, fine di limitare privilegi - ammesso che vi siano - ma per escluderli e stabilire, invece, che quanto ci compete ci spetta per la dignità di rappresentanza del popolo italiano.

un'Aula parlamentare chieda al Governo di sostituirla nell'iniziativa legislativa. Non si è mai visto che un collega senatore chieda al Governo di presentare un emendamento invece di ricorrere ad una sua iniziativa parlamentare.

Io rivendico all'iniziativa parlamentare il primario potere legislativo e ritengo inammissibile che noi stessi ci si spogli di questo potere e si chieda al Governo di sostituirci nell'iniziativa legislativa. Presidente, chiedo - lo ripeto

esaminando una Nota di variazioni al DPEF che parla della vita degli italiani e del Paese, ma parliamo di queste cose, pure importanti.

procedere alla votazione dell'emendamento, poiché poco fa sono state sollevate alcune eccezioni circa la possibile ammissibilità di questi due emendamenti, vorrei semplicemente ricordare, a coloro che hanno manifestato un'opinione diversa dalla Presidenza, che quando il 17 luglio 2006, con il decreto n. 233, il Governo attualmente in carica aumentava il numero dei Ministri, prevedeva una norma di copertura della spesa da ciò derivante. Voglio anche ricordare che nella legge finanziaria presentata oggi da questo Governo, nella relazione che fa riferimento all'articolo 14, si legge che viene inoltre prevista, in un'ottica del contenimento della rappresentanza, la riduzione del numero dei consiglieri comunali. Tant'è vero che questa norma è prevista e specificata sempre nell'articolo 14, esattamente al comma 2. Mi domando: se è regolamentare, se è confacente al rispetto delle leggi vigenti la norma presentata dal Governo, che ha sicuramente un carattere ordinamentale perché cambia il numero dei consiglieri comunali, perché non devo avere un carattere ordinamentale e non essere quindi rispettoso delle prerogative dell'*iter* del Parlamento un emendamento che interviene praticamente su una materia che è sia di spesa, sia anche ordinamentale. Per questa semplice ragione abbiamo accolto gli emendamenti che sono stati presentati: diversamente, senatore Morando, la Commissione che lei presiede avrebbe dovuto esprimere un parere contrario all'articolo 14, terzo

grazie.

Signor Presidente, anch'io intervengo solo per annunciare il voto favorevole alla risoluzione firmata dal collega Vegas, da me e da altri di prestarmi un minimo di attenzione, per tre secondi. Ho letto una Nota di variazione al DPEF nella quale il Governo propone (e voi lo state votando)... Nella Nota di variazione al DPEF stampata è scritto che il Governo aumenta il *deficit* pubblico, riduce l'avanzo primario, aumenta il debito pubblico, aumenta la pressione fiscale e la spesa pubblica: è scritto nelle tabelle della versione

dal Governo e da questa maggioranza. Questo è scritto negli andamenti tendenziali rispetto a quelli programmatici. Per questo motivo, denunciando la schizofrenia di questo Governo e di questa maggioranza, voteremo «no» alla risoluzione della maggioranza.*(Applausi

Grazie

di riferire a quest'Aula di presunti falsi in bilancio: lui se ne intende, con gli altri suoi colleghi dell'opposizione, di falso in bilancio, essendosene occupato ampiamente, con gli esiti che conosciamo, dal Gruppo FI)*. La verità è un'altra: nel passato, tutte le previsioni economiche e finanziarie si sono rivelate errate, come ampiamente dimostrato, e invece quest'anno, con la manovra economica che che esamineremo prossimamente si dimostrerà - e lo si fa anche con la Nota di aggiornamento al DPEF - che le previsioni sono state tutte azzeccate

ma faccio notare, soltanto affinché venga messo agli atti, che il mio riferimento è preciso e puntuale alle tabelle pubblicate nella Nota di aggiornamento trasmessaci dal Governo. gli andamenti tendenziali (cioè se non si facesse nulla) del *deficit* pubblico, dell'avanzo primario e del debito pubblico sarebbero più bassi dopo l'intervento del Governo. Ciò vuol dire che, secondo queste tabelle, la maggioranza consapevolmente o inconsapevolmente ha delegato il Governo ad aumentare il *deficit* pubblico, ad aumentare il debito pubblico, a ridurre l'avanzo primario, ad aumentare la pressione fiscale ed anche la spesa pubblica. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con quanto ha affermato il collega Legnini. Non si tratta di un discorso di previsioni: non c'entra nulla! L'andamento tendenziale è stato dichiarato dal Governo: rispetto a quell'andamento, l'Esecutivo propone di sfasciare la finanza pubblica aumentando *deficit* e debito pubblico. signor Presidente, del quadro macroeconomico degli andamenti di crescita che determinano ulteriori rischi sul risanamento finanziario del Paese. Quindi, avete approvato un indirizzo al Governo per concedere allo stesso Governo la possibilità di frenare la crescita, di aumentare il *deficit* pubblico, la spesa pubblica ed il debito pubblico rispetto - ripeto - agli andamenti

Le chiedo, signor Presidente, di intervenire sollecitamente perché riguarda i risparmi sugli interventi energetici previsti nella legge finanziaria 2007,

Padoa-Schioppa, però, nell'illustrazione dell'altro giorno, ha riproposto i medesimi interventi per la finanziaria corrente. Credo, quindi, sia da chiarire se i cittadini possono beneficiare di tali interventi perché quelli che hanno eseguito i lavori per l'anno corrente

in piena legittimità considerata invece improponibile da lei e dalla Presidenza, è di significativo rilievo per lo sviluppo immediato dei nostri lavori. inutilizzabile l'argomento che fa riferimento al contenuto dell'attuale disegno di legge finanziaria depositato dal Governo in Senato per sostenere che, poiché lì vi sono norme meramente ordinamentali,

Oggi pomeriggio, quando il Senato riprenderà i suoi lavori, il Presidente del Senato, sulla base di un'attività di consulenza svolta dalla Commissione Bilancio,

nel disegno di legge finanziaria di norme meramente ordinamentali che, come tali, violano la legge di contabilità. Tale provvedimento dice chiaramente che la legge finanziaria non prive di effetto finanziario aventi carattere meramente ordinamentali perché quelle norme, quando riguardano lo sviluppo dell'economia, devono essere contenute nei disegni di legge collegati che si discutono fuori dalla sessione di bilancio.

esaminato ieri dalla Commissione bilancio in sede di dibattito per la formulazione del parere al Presidente per la sua delibera sul contenuto proprio, sono state fatte oggetto di indagine e analisi da parte della Commissione Bilancio. Le posso anticipare che una quantità molto significativa di queste norme, più di quanto non sia accaduto gli anni scorsi, sarà oggetto di proposta di stralcio.

intanto sarebbe da considerarsi ammissibile in quanto il disegno di legge del Governo conterrebbe norme dello stesso carattere. Non nego che sia così ma esattamente su quelle norme aventi quel carattere la Presidenza del Senato dovrebbe, a mio parere, pronunciarsi con una deliberazione di stralcio. In ogni caso, ciò proporrà la Commissione Bilancio. Quindi, sotto il profilo sistematico e per l'ordine dei nostri lavori, bisognerebbe considerare che la Presidenza ha preso

1, comma 25, si fa riferimento all'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, Vice ministri, Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi 1, 8 e 19 dell'articolo 1, che istituisce

l'intervento di carattere ordinamentale con la giustificazione di una riduzione dei costi di spesa. Questa è l'interpretazione che abbiamo dato allo stato dell'arte. Attendiamo questa sera, non volevo assolutamente né invadere il campo della Commissione che lei presiede, né, tantomeno, anticipare il giudizio che sulla finanziaria darà il Presidente del Senato. Staremo a vedere: hanno seguito più e meglio di me, con maggior competenza di me, queste questioni, vedremo e valuteremo, e poi ne discuteremo nel merito, nelle prossime settimane. Grazie comunque, senatore Morando, per il contributo.

Presidente, volevo richiamare la sua attenzione sulle notizie di stampa di questa mattina e, in particolare, sul servizio molto documentato e assai inquietante del quotidiano di Torino «la Stampa» firmato, tra l'altro, da un giornalista che solitamente è molto informato e non è sospetto di particolari pregiudiziali nei confronti della magistratura, anzi tutt'altro. Pare che un magistrato della Procura della Repubblica di Catanzaro, da un po' di tempo, raccolga, scavalcando il Ministero dell'interno e delle comunicazioni e i loro servizi e rivolgendosi direttamente ai gestori delle telefonie, i tabulati delle conversazioni telefoniche di mezza Italia, ivi compresi i tabulati delle conversazioni del Presidente del Senato, del Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e anche di molti suoi colleghi magistrati. cioè, creato un archivio, in una stanza dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che non avrebbe niente da invidiare ai famosi archivi del SIFAR del generale De Lorenzo. Perché questo magistrato abbia fatto e faccia questo non si sa, anche se non è difficile immaginarlo. Io credo che sia il caso che il Governo si interessi rapidamente a questa questione e venga a riferire in Grazie, senatore Iannuzzi, riferiremo immediatamente di questa sua segnalazione. Suppongo che sarà stata rivolta anche all'attenzione del Ministro competente, ma penso che dovremmo rivolgere la medesima

perché non può che destare grande inquietudine ciò che abbiamo letto oggi sui giornali. Io mi chiedo a che titolo questo magistrato abbia acquisito tali dati, *contra legem*, questo è bene sottolinearlo, signor Presidente, perché non si sono seguite le procedure consuete in forza delle quali si può avere accesso a questa documentazione tutta particolare. Con criteri assolutamente arbitrari si è costituito questa sorta di *database*, questa banca dati dove ci sono i numeri di telefono di autorevoli esponenti della Repubblica. Per quale ragione? Per quale motivo? Cosa c'entra tutto questo con le indagini in corso? Io ho l'impressione che tutto questo serva ad alimentare la confusione e a vanificare gli esiti delle indagini. Se non fosse già sufficiente, per ipotizzare un risultato di questo genere, bisognerebbe conoscere le pronunzie giurisdizionali che ogni volta hanno infranto in maniera sistematica tutte le iniziative avviate da questo magistrato nell'ambito dei processi dei quali oggi la stampa,

anche perché la sua utenza, sulla base delle cose che abbiamo letto, è stata acquisita, cioè il suo numero di telefono è stato acquisito nel novero di questi tabulati che dovevano servire non si sa bene a cosa

Trovo che francamente sia invincibile il sospetto che ben altre ragioni siano sottese a questo atto così clamorosamente illegittimo. Credo che il Senato e il Governo debbano intervenire e mi auguro che in tempi brevi si possa capire ciò che sta accadendo. Voglio concludere ricordando che c'è un'area della politica, devo dire residuale, che in questo momento sta agitando le piazze contro le legittime iniziative che sono state avviate nei confronti di questo magistrato. Questo è un fatto molto grave e forse l'acquisizione

Bivona, Porto Salvo e Longobardi, aree importanti, assumeva la forza e la violenza di una vera e propria alluvione, distruggendo immobili e beni privati dell'intera popolazione dei centri summenzionati, causando diverse vittime, sei morti, e oltre 50 feriti. oltre 50 feriti. Forse qualcuno saprà che l'intero sistema turistico, forse l'unica fonte di sostentamento per molte famiglie dipendenti di aziende del settore stesso e di altri settori contingenti, nonché le varie piccole e medie imprese che hanno sede nelle zone colpite, subirono ingentissimi danni, tali da costringere oltre 2.000 lavoratori a divenire disoccupati ed entrare in una fase di forte disagio e di miseria assoluta. Signor Presidente, qualcuno forse ricorderà che nella legge finanziaria per il 2007 erano previste delle somme di denaro - per la verità nemmeno ingenti, con ogni probabilità nemmeno bastanti a dare risposta ai gravissimi danni e ai gravissimi problemi problemi della popolazione - ripartite in tre anni, da destinare alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio colpito dalla calamità naturale. Forse però davvero non si sa che a distanza ormai di 15 mesi non si ha ancora nessuna notizia dei fondi stanziati dal Governo, né se essi sono stati erogati, né di chi li debba gestire. La popolazione a Vibo Valentia così come in tante altre aree della Calabria, per la verità, si è costituita in comitati civici in difesa dei propri diritti e lamenta uno stato di drammatico abbandono da parte delle autorità. Tali comitati sono pronti anche a forme di lotta particolarmente forti e significative, sino a giungere anche a protestare di fronte al Senato. La maggior parte della popolazione delle zone colpite denuncia di non aver avuto ancora il risarcimento per i danni subiti. Vi sono molti casi in questi giorni di cittadini che per poter ristrutturare la propria abitazione e riprendere la loro vita normale sono costretti a ricorrere a mutui e a prestiti finanziari, in mancanza

Non vorrei che di nuovo Cristo si fermasse a Eboli o che lì, a Melfi, o a Mirafiori si fermasse anche il Governo Prodi e l'intero centro-sinistra.

Avevo lasciato cadere l'argomento che trattava il testo dell'interrogazione riguardante il ritardo il quale fu possibile mettere in funzione l'autoambulanza nella quale io fui ricoverato per fibrillazioni cardiache. L'avevo lasciato cadere perché pensavo che le polemiche politiche si esaurissero, ma oggi si è aggiunto invece il fatto che devo rispondere in sede penale di due reati, precisamente interruzione di pubblico servizio e truffa aggravata. Vorrei quindi conoscere gli elementi che possono venire dalla risposta che il Governo penso dovrà dare.

di fare la cavia del non funzionamento del servizio, che doveva essere di massima rapidità.

il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto opportuno agire e il mio caso giudiziario è passato subito al giudice dell'udienza preliminare. Quindi, sarebbe urgente una risposta alla mia interrogazione per vedere come viene considerato dal Governo il disservizio che ho dovuto lamentare

sulla casa circondariale di Crotone, riguarda il lavoro straordinario ed il contenzioso che contrappone gli agenti di polizia penitenziaria e la locale amministrazione del carcere. La seconda interrogazione questione è più importante sul piano nazionale, avendo avuto anche attenzione mediatica.

quale, esattamente come nel caso del senatore Selva, mi trovo nella condizione di dover rispondere alla giustizia. Voglio capire quante volte è stato applicato. Ho sollecitato

legge quello di Grillo, che cancella quelli che sono contro di lui, stante la notizia di ieri della polizia postale. Non le dico, signor Ministro, cosa dovrei chiedere per tutti quelli che scrivono "Storace, ti odio"; lei ha un potere che riesce ad esercitare e le faccio i miei complimenti.

volontà di rispondere al Parlamento e allora, presidente Angius, vorrei sapere: questa barzelletta dei solleciti la dobbiamo considerare tale o c'è speranza che il Senato faccia sentire la sua voce ai Ministri che non vogliono rispondere? Non è una barzelletta, senatore Storace. La Presidenza del Senato il sollecito lo fa immediatamente. La responsabilità della risposta non compete però, nonostante la sollecitazione tempestiva, alla Presidenza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto esterrefatto nel leggere oggi su «la Stampa» di Torino un servizio, a firma Guido Ruotolo,

riguarda anche i vertici dello Stato e delle istituzioni, pezzi della magistratura, le forze di polizia, parlamentari ai vertici delle istituzioni del Paese, in un intreccio inquietante e fosco di trame che hanno molto di eversivo e di anticostituzionale. Quando si attenta al privato delle utenze delle massime cariche dello Stato e si mette in moto un meccanismo di permanente e sistematica delegittimazione, con la ricerca di numeri telefonici, senza un minimo di procedura regolamentare, la questione inquieta e preoccupa. Per queste ragioni e per le ragioni che sono state chiaramente espresse dai senatori Iannuzzi e Valentino, chiediamo che il Presidente del Consiglio dei ministri venga a riferire in Aula, per liberare il campo da queste incursioni che avvengono in alcuni uffici giudiziari italiani e che confermano il clima che vive il Paese, un clima di antipolitica, un clima corrosivo,

per la sua presenza fino alla fine della seduta - sulla vicenda del terrorista in trasferta a Siena, che godeva dei benefici premiali della legge Gozzini. Riteniamo debba essere data una risposta urgente a tale questione, considerata la sua delicatezza, perché viene offesa la memoria di tante vittime del terrorismo, in particolare la famiglia Berardi, colpita profondamente. È una questione che colpisce l'opinione pubblica. Bisogna chiarire l'intreccio tra cooperative sociali e amministrazioni comunali. Bisogna capire se vengono fatti controlli su questi ex terroristi, che ottengono case e trovano impiego con grande facilità, cosa che non è permessa evidentemente alle persone normali, e se durante le ore di lavoro per i benefici premiali

delle dichiarazioni del suo sottosegretario Manconi, il quale ha affermato che la legge Gozzini funziona bene. La legge Gozzini non funziona bene se pluricondannati all'ergastolo si trovano nelle condizioni di poter compiere reati così gravi.

il professor Giovanni Sartori, non ho ben compreso - appunto perché mi è stato riferito - se in relazione all'attuale o alla precedente legge elettorale, sostanzialmente affermato che tutti i parlamentari, da Roma in giù, praticamente sono stati eletti con i voti mafiosi o criminali. Credo che se questa affermazione è vera

se questa affermazione rientra nella legittima valutazione sul funzionamento e sull'impatto dei sistemi elettorali è un conto; ma poiché, a volte, in trasmissioni televisive

di tanti dibattiti e di tante discussioni sulla delegittimazione della rappresentanza popolare. Signor Presidente, la invito a verificare e, se del caso, ad assumere tutte le iniziative per tutelare la dignità del Parlamento e dei parlamentari, soprattutto dei parlamentari meridionali. Senatore Viespoli, su quest'ultima sua sollecitazione francamente possiamo verificare, ma è difficile intervenire. Capisco che "Porta a Porta" è considerata ormai la terza Camera; è difficile però che il Senato e la sua Presidenza possano intervenire circa le dichiarazioni del professor Sartori, al quale al massimo possiamo concedere le attenuanti generiche per quanto ha Naturalmente sarà compito nostro difendere la dignità del Senato, come lei ha precisato, e dei senatori eletti a Sud di Roma (ma anche di quelli eletti a Nord di Roma).

dai diversi colleghi, per primo dal collega Iannuzzi e successivamente da altri, circa un articolo di stampa, pubblicato sul quotidiano "la Stampa", quale si dà notizia dell'acquisizione di migliaia di tabulati telefonici di cittadini da parte del sostituto procuratore di Catanzaro, Luigi De Magistris, moltissimi quali riguarderebbero personalità istituzionali e politiche, tra cui magistrati, vertici della Polizia di Stato, vertici di Governo e delle istituzioni, che sarebbero stati oggetto appunto di tale intervento da parte del magistrato, con una conseguente conservazione dei tabulati telefonici, la Presidenza del Senato giudica tale notizia di estrema gravità. al Ministro della giustizia e al Ministro dell'interno dell'estrema urgenza, che qui è stata giustamente richiamata, di rispondere alle interrogazioni ed alle interpellanze che su tale questione, proprio nella giornata di oggi, sono già state depositate presso gli Uffici del Senato da diversi colleghi di entrambi gli schieramenti. Sarà pertanto compito nostro procedere in questo senso e in questa direzione.

La seduta è tolta